Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle deleghe di funzioni conferite dai Ministri dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, è stato attribuito il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

I colleghi ricorderanno che il 1° agosto in quella sede c'è stata una votazione sulla candidatura espressa dal consiglio di amministrazione e sottoposta al voto in Commissione di vigilanza sul presidente candidato Marcello Foa. Quella votazione ebbe esito negativo. Il Partito Democratico riteneva e ritiene ancora oggi che con quella votazione la candidatura del presidente Marcello Foa non potesse essere ripresentata. Nonostante questo, dopo due mesi di blocco dell'attività della più grande azienda culturale pubblica (e due mesi sono tanti, signor Presidente),

ad una votazione illegittima su una candidatura illegittima. Questa seduta della Commissione di vigilanza ha avuto luogo il 26 settembre,

Si è votato, ma evidentemente l'accordo che fu fatto a cena con il presidente Berlusconi, da parte del ministro Salvini in rappresentanza anche del MoVimento 5 Stelle, aveva

alla fine dello spoglio sono appena sufficienti per l'elezione, sono giusto quelli necessari, ma questo non è il dato reale di tale votazione. Questo non corrisponde a quanto è successo nelle urne. Per le informazioni che abbiamo ricevuto per le vie brevi, per le vie brevi, riteniamo che all'interno del seggio ci sia stata una forzatura interpretativa: riteniamo che due di queste 27 schede fossero da annullare, anzi, riteniamo che i votanti di queste due schede abbiano votato in un certo modo proprio perché volevano, desideravano che quelle schede fossero annullate. Quindi, in realtà, i voti validi in quella seduta furono 25 e il presidente Foa, nonostante non avesse neanche il diritto di essere nuovamente candidato, non può essere eletto come presidente della RAI. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Allora noi abbiamo chiesto semplicemente al presidente Barachini, già a conclusione di quella difficile giornata, di avere accesso agli atti per verificare queste schede. Poi le valutazioni, l'autorevolezza e l'autorità del presidente Barachini, rispetto al merito, rimarranno tali comunque. Lui ha negato l'accesso agli atti. Certamente, si è ispirato, con una sua interpretazione, al Regolamento, però su un fatto e su una nomina così importante non è accettabile, da parte

questa parola da questa bruttissima vicenda: verificare le schede e capiremo se i brogli ci sono. con riferimento a tale lettera e alle osservazioni che oggi ha svolto in Aula, voglio rassicurarla che, nelle forme che saranno proprie, avrò modo di fornirle tutti i chiarimenti che lei ha richiesto.

sugli sviluppi della situazione in Libia». Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, professor Moavero Milanesi. Signor Presidente, senatrici e senatori, mi scuso perché, come adesso anticipava il Presidente, dovrò andar via dopo il mio intervento. Iniziava più o meno in orario corrispondente a questa presentazione questa presentazione in Aula una riunione di Ministri (non è proprio un Consiglio dei ministri, ma una riunione sulle questioni economiche), come peraltro annunciato anche da alcune agenzie giornalistiche. Mi dovrò recare in tale sede però tenevo a mantenere doverosamente l'impegno nei confronti dell'Assemblea, com'era stato richiesto,

Brevemente, per punti schematici, cerco di riassumervi la situazione. Nelle ultime settimane ci sono state una serie di sviluppi che hanno investito sia la sicurezza della già tribolata situazione in Libia, sia gli aspetti di carattere economico. Sono state anche settimane - parlo dell'ultimo mese e mezzo - caratterizzate da una serie di intensi contatti

in primo luogo, ai rappresentanti del Governo riconosciuto dalla comunità internazionale, il presidente Sarraj e il ministro degli esteri Siala, e all'inviato dell'ONU Salamé. Penso anche al vice presidente Maitig, che è venuto di recente a Roma e con il quale abbiamo frequenti rapporti. Io mi sono anche recato - come penso già sappiate - in Cirenaica, a Bengasi, a incontrare il maresciallo di campo Haftar.

di molti *leader* internazionali a New York per la settimana dell'ONU. Credo che i principi ai quali ci stiamo attenendo sullo scenario libico siano a voi siano a voi tutti noti, ma utili da riprendere e ricordare. Il primo riguarda il pieno riconoscimento da parte nostra, come Italia, della necessità di un'assunzione di responsabilità da parte dei protagonisti dello scenario libico, delle istituzioni

che è giusto che il popolo e le istituzioni di uno Stato abbiano sulla loro realtà e sul loro futuro. Questo è il primo grande principio. Il secondo principio a cui ci atteniamo è quello del dialogo con tutti gli interlocutori affidabili dello scenario libico e *in primis* con i rappresentanti del del Governo riconosciuto dalla comunità internazionale. Anche quest'ultima cosa sembra ovvia, è relativamente ovvia in una situazione difficile, ma è importante ricordarla, perché, come Italia, dobbiamo sempre muoverci in un contesto di principi di diritto internazionale nel quale ci siamo sempre riconosciuti, in particolare nel corso terzo principio è quello della centralità delle Nazioni Unite. Esiste una missione speciale dell'ONU, con un rappresentante speciale, il libanese Salamé, che opera nello scenario libico e che ha preparato un piano, un percorso delle varie cose da fare che si accinge anche a rivedere. Il signor Salamé si trova a Tripoli e segnalo che vi è rimasto anche durante la settimana dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, proprio come segnale nei confronti della popolazione civile della presenza del delegato ONU, un segnale che credo comprendiamo tutti sia percepito come rassicurante. Stiamo parlando quindi di una persona che non solo è dotata di un incarico molto importante e cruciale, ma è e opera sul terreno. altro principio a cui ci atteniamo è quello della necessità di garantire quanta più coesione possibile nell'ambito dei rapporti tra la comunità internazionale, gli Stati della comunità internazionale (quindi tutti i vari Stati del mondo) e la Libia. Anche qui, sembra che siano tutte cose evidenti, ma teniamo conto - credo non sfugga a nessuno in quest'Aula quest'Aula - che questi Stati, che magari sono tutti collaboranti e anche pieni di buone intenzioni per un processo di pace e stabilizzazione, poi si fanno una certa competizione, ad esempio, sul piano dell'influenza economica (per citare quello più frequente). Quindi, bisogna mantenere un rapporto tale da permettere a questa miscela di cooperazione e competizione di operare al meglio e non a danno degli interessi della Libia e del suo popolo. Ricordo poi l'importanza del rafforzamento del nostro rapporto bilaterale con la Libia, che ci è stato più parti e da tutte le parti dello scenario libico da me incontrate. Diciamola pure così: c'è un'apertura e un desiderio di presenza italiana, vista come una presenza che può facilitare. Naturalmente, c'è poi la normale reazione di diffidenza quando certe presenze (eventualmente anche la nostra) possano essere percepite, da questa o da quest'altra parte, come antitetiche; in uno scenario così in movimento, è più che normale.

dal punto di vista della sicurezza, proprio della sicurezza materiale, quella a cui noi, in Paesi più normali, siamo totalmente abituati. Sul piano della sicurezza materiale, abbiamo visto le recrudescenze di conflitti armati, abbiamo visto vari cessate il fuoco, accordi di tregua e quant'altro. È una situazione che presenta punte di criticità, soprattutto nell'area della città di Tripoli, area in cui peraltro è concentrata buona parte della popolazione urbana e della popolazione della stessa Libia. Rispetto a questo noi come Italia, siamo totalmente a supporto degli degli sforzi delle Nazioni Unite e quant'altro per la tregua e per il consolidamento della medesima. Come ogni tregua, anche questa ogni tanto viene interrotta; ci auguriamo che gli ultimi accordi raggiunti il 23 settembre riescano ad avere una tenuta di durata superiore, ma la situazione resta fragile ed è anche importante garantire che l'uscita dall'area urbana di Tripoli di determinate milizie, che non facevano parte di quel territorio come origine abituale, sia e diventi abituale, sia e diventi un acquisito permanente, in modo che la cessazione delle ostilità possa consolidarsi e che gli accordi per la sicurezza della capitale libica possano essere pienamente applicati e diventare pienamente funzionali. Questo non solo dal punto di vista del di vista del principio stesso e dell'importanza materiale della sicurezza, ma anche perché - non dimentichiamolo mai - quando ci sono questi scontri armati, oltre a esserci vittime tra le milizie e le truppe combattenti, ci sono numerosi atti di violenza materiale sulle popolazioni civili, che sono poi la parte a cui dobbiamo prestare più attenzione dal punto di vista della civiltà dei diritti fondamentali e dei principi umanitari che ci sono propri, anche come posizione italiana. Il quarto elemento alla vostra attenzione è quello relativo agli sviluppi politici interni in Libia. Come sapete, negli accordi che erano stati stipulati in occasione degli incontri a Parigi qualche mese fa era stata molto focalizzata l'idea non solo di avere delle elezioni, che sono il momento culminante di un processo di stabilizzazione democratica di qualunque Paese e popolo, ma soprattutto di stabilire data delle elezioni, che era stata fissata al 10 dicembre e sostanzialmente concordata, o comunque non negata, dalle parti che erano state convenute a Parigi. Rispetto a questa data, la nostra posizione, come Italia e come Governo italiano, è sempre stata che naturalmente vedevamo le elezioni come un momento indispensabile ma, proprio in quanto momento indispensabile e coronamento di un processo democratico che chiama un popolo a esprimersi sulle sue istituzioni ritenevamo che queste dovessero svolgersi in condizioni costituzionali e legislative chiare e in condizioni di piena legittimità, credibilità e trasparenza, per avere in questo modo l'effetto auspicato. Per cui per noi poteva essere il 10 dicembre, ma anche il 9, l'11 o o più probabilmente un'altra data; non era importante la questione della data, ma era importante che ci si arrivasse nelle condizioni migliori. Fra le condizioni, era indispensabile che il Parlamento libico, che si riunisce nella città di Tobruk, si esprimesse sul quadro costituzionale (questo richiedeva anche un passaggio referendario) e che emanasse una legge elettorale in base alla quale si sarebbero tenute le elezioni. Sono andate a vuoto varie sedute, malgrado i preannunci del Parlamento libico, e soltanto ultimamente è stato trovato un accordo, in condizioni di voto in parte contestate, perché il *quorum* è stato raggiunto attraverso firme raccolte anche fra chi non era presente (insomma una situazione complessa). In ogni modo, ci sarebbero le prime condizioni base, ma solo recentissimamente. Noi pensiamo che su questo si debba costruire il resto del percorso. Naturalmente, ripeto, nessuno ha mai messo in dubbio da parte del Governo italiano e, mi permetterei di dire, da parte italiana, che si debbano tenere le elezioni, ma riteniamo che si debbano tenere nelle condizioni

Il quinto elemento che vorrei portare alla vostra attenzione riguarda le questioni legate all'economia della Libia, che si regge molto anche sull'estrazione di idrocarburi. Il Paese ha un'economia con delle potenzialità importanti che però sono state messe ampiamente in crisi dalla situazione conflittuale che esiste oramai da molto tempo. Per noi è sempre stato essenziale - e la posizione del Governo italiano è sempre stata molto chiara al riguardo - che le istituzioni centrali unitarie della Libia, in particolare la Banca centrale per la parte per la parte economico-finanziaria e la Compagnia nazionale degli idrocarburi, la cosiddetta NOC, rimanessero istituzioni centrali unite unite con la piena approvazione e la garanzia dell'ONU. Su questo punto siamo impegnati. Siamo anche impegnati al sostegno di un pacchetto di riforme che è stato adottato il 12 settembre dal Consiglio presidenziale e fatto proprio, poi, dall'Alto consiglio di Stato, la Camera alta della Libia, se vogliamo vederla in una tipologia di schema costituzionale a noi più familiare, e dalla Banca centrale. Questo pacchetto di riforme ricomprende, in particolare, quattro elementi: una tariffa di acquisto della valuta estera per riallineare il tasso di cambio (questione importante in Libia come altrove, al fine di mantenere tariffe di acquisto di valuta estera corrette); riduzione delle sovvenzioni governative sul carburante; l'aumento di 1.000 dollari dell'indennità governativa annuale a favore delle famiglie libiche (possiamo ben renderci conto della situazione in cui versa molta parte della popolazione civile); l'incremento dei contributi per le spese mediche e universitarie. Si che fanno parte di tentativi di riforma essenziali per avvicinare le situazioni della Libia, quanto più possibile, alla normalità. Quindi anche l'aspetto delle riforme economiche, raccomandate peraltro dalle Nazioni Unite e dal contesto della comunità internazionale, è molto importante per riportare situazioni corrette in Libia, che fanno parte del processo definibile di normalizzazione sesto elemento è il processo politico internazionale. Abbiamo avuto elementi importanti da vari incontri, in particolare, come vi dicevo, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite la settimana scorsa, nella quale si sono svolte anche una serie di riunioni dedicate alla Libia, con la partecipazione in videoconferenza dell'inviato ONU Salamè. Ho avuto incontri bilaterali con i Ministri degli esteri di Francia, Emirati Arabi, Qatar, Marocco, Egitto, con il Segretario Generale della Lega araba e

sostanziale volontà di lavorare per la soluzione, pur esistendo fra alcuni degli interlocutori che vi ho appena nominato, delle diversità di vedute. Se dovessi setacciare quanto raccolto, vedrei cinque punti di comune denominatore. Il primo è che tutti si esprimono a favore di un'assistenza, di un sostegno, di un supporto all'azione del delegato ONU Salamè. È importante, perché se lui ha il riconoscimento delle varie parti in causa, può portare avanti al meglio il processo. Il secondo punto è l'essenzialità di riportare la sicurezza a Tripoli, che vuol dire la fine degli scontri armati, il mantenimento della tregua Il terzo punto di comune denominatore è di mantenere viva la prospettiva delle elezioni. Ripeto: anche se la data del 10 dicembre, come appare alquanto ineluttabile, non dovesse essere rispettata, ciò non vuol dire affatto che le elezioni stiano tramontando o stiano andando "in dissolvenza", per usare un termine della fotografia di un tempo. In realtà, l'idea delle elezioni deve rimanere un punto fermo, perché è lì che

fra loro dinamicamente conflittuali. C'è dialettica (nessuno lo nega e probabilmente è anche bene che ci sia dialettica, perché nessuno può pretendere di avere il monopolio della soluzione o della ragione), ma questa dialettica non è

rivalità accesa e conflittuale (in senso pacifico, ma pur sempre di contrapposizione) fra noi e i francesi.

con il presidente Trump, che esiste una volontà americana di appoggiare l'azione italiana nell'ambito dello scenario libico e, in maniera più vasta, nell'ambito del Mediterraneo: su questo possiamo possiamo contare. Tra l'altro, segnalo che anche oggi, nel corso di riunioni NATO a Bruxelles, è stato confermato l'impegno a un riorientamento dell'Alleanza atlantica verso il suo fianco Sud, il che vuol dire Mediterraneo e maggiore attenzione a un'area geografica cui noi rivolgiamo, per ragioni

tutti gli altri, della Conferenza per la Libia, della quale vi fornisco alcuni elementi ulteriori. Il programma è tenere una Conferenza

attenta a ciò che accade sull'altra sponda del Mediterraneo. In questo senso teniamo anche a sottolineare quello che prima vi dicevo con un gioco di parole, ovvero che la Conferenza è «per la Libia», e non «sulla Libia» nella capitale di uno Stato che ritiene di avere chissà quale ricetta miracolosa per risolvere i problemi, proprio per cercare di facilitare. L'obiettivo è quindi facilitare il processo di securizzazione in Libia. Saranno invitati i principali interlocutori dello scenario libico, a cominciare naturalmente da quelli che ho già nominato e che ho già incontrato: *in primis*, il Governo riconosciuto dalla comunità internazionale. Abbiamo avuto conferma anche ieri dell'interesse e della presenza del maresciallo di campo Haftar e ci saranno naturalmente anche altri interlocutori del complesso scenario. Inviteremo i Paesi vicini confinanti, i Paesi vicini per affinità di popolazioni. Inviteremo i Paesi europei maggiormente interessati a quanto accade in Libia; inviteremo, naturalmente, i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: Stati Uniti, Cina, Russia, oltre agli altri due membri europei che

che si trova ad avere un interesse geopolitico, o più eminentemente di ruolo internazionale, allo scenario libico. L'obiettivo è facilitare il dialogo: sembra un obiettivo minimale ma in realtà, quando pensate gli scontri armati a Tripoli, non lo è. Vorremmo rimanere all'interno del principio della completa autodeterminazione libica, che è evidentemente un punto fondamentale, una loro presa di di responsabilità; è anche estremamente importante che ci sia un approccio inclusivo. L'obiettivo è identificare le tappe del processo di stabilizzazione. In questo caso, in particolare, qualora fosse ulteriormente verosimile che non si potranno tenere le elezioni alla data immaginata, vorremmo evitare di stabilire altre date, ma evidenziare le varie tappe che andranno seguite per arrivare al momento fondamentale delle elezioni. Quindi, non sarà una Conferenza che impone scadenze o che detta compiti, quanto una Conferenza in cui i diretti interessati si potranno dare un'agenda comune e identificare i passaggi. Infine, l'ultimo punto che vorrei toccare con voi riguarda l'operatività della nostra ambasciata a Tripoli. Sapete che siamo fra i pochi Paesi ad avere un'ambasciata aperta a Tripoli, e la nostra ambasciata è ed è rimasta sempre operativa, anche se, per motivi di sicurezza, durante il periodo degli scontri, come avviene generalmente in questi casi, abbiamo ridotto il personale. È comunque presente, oltre a personale militare per motivi di sicurezza, anche personale civile che svolge le normali pratiche dell'ambasciata. Il Il periodo di recrudescenza degli scontri nell'area di Tripoli era stato preceduto da una situazione non ideale, per quanto riguarda la persona del nostro ambasciatore a Tripoli, che aveva fatto seguito a un'intervista

sia a livello di presa di posizione da parte dei diversi interlocutori delle varie autorità libiche. Tengo a precisare che queste prese di posizione critiche sono state manifestate da tutti gli interlocutori dello scenario con cui abbiamo avuto contatti, a cominciare (come primi a reagire) dalle autorità del Governo riconosciuto dalla comunità internazionale: il presidente Sarraj, il Ministro degli esteri e gli altri interlocutori. A seguito di ciò, essendo stati espressi dei dubbi, confermati

ancora attualmente. Naturalmente questa non è una situazione positiva in un momento in cui avremmo la necessità di essere pienamente operativi, ma si è venuta a determinare e abbiamo dovuto prenderne atto. Ad ogni modo, ripeto, l'ambasciata è operativa e la Conferenza si terrà. In particolare, il vice ministro Emanuela Del Re, ora presente in Aula (che mi sostituirà quando purtroppo dovrò andare via), collaborerà strettamente nell'organizzazione

utile a voi per ulteriori riflessioni. Ribadisco davanti all'Assemblea e a lei, signor Presidente, il mio impegno personale, come Ministro della Repubblica, a riferire regolarmente in Aula, se necessario, e nelle Commissioni parlamentari; questo vale nei confronti di questo come dell'altro ramo del Parlamento, nei confronti del quale mantengo

Signor Presidente, francamente non è semplicissimo intervenire adesso. Abbiamo sentito da parte del sempre cortese e

Il Ministro, alla fine, ha lasciato cadere con diplomazia una frase: ha parlato con il suo collega francese, con cui, come voi sapete, abbiamo

di cosa stiamo parlando? Stiamo avviandoci verso la Conferenza di Palermo, ma quello che purtroppo drammaticamente - perché non si può minimizzare ci viene detto oggi è che tra italiani e francesi su questo*dossier* c'è ancora una visione completamente diversa. Se devo decrittare la formalità e la diplomazia, sempre amabile, del ministro Moavero Milanesi, traggo la deduzione che i francesi, che in questi anni hanno remato in una direzione opposta, *pro*-Haftar, insieme a Egitto e ad altri attori ragionali,

di Palermo uno è così stanco che non può più continuare, ci sono tutti. Scusate colleghi, ma la politica internazionale si fa per le celebrazioni, per la retorica, per le affermazioni di volontà generiche e si fa per i risultati. Andiamo a una Conferenza e adesso abbiamo saputo che tra gli attori principali di questa vicenda,

che stiamo amministrando da anni e in cui da anni constatiamo che ci sono diverse parti in commedia, che non sono accettabili. Il fatto che i due principali attori della

(comunque sbagliata, visto l'effetto), egli è dovuto riparare rapidamente in Italia. Parteciperà all'elaborazione dei documenti della Conferenza di Palermo, ma è meglio che non torni in Libia, perché tutti gli attori

è veramente inaccettabile. Stimo questo diplomatico, l'ho conosciuto e credo che sia un diplomatico valente, ma non può rimanere alla testa di un'ambasciata aperta senza di lui: l'ambasciatore sta a Roma e l'ambasciata è aperta e pienamente operativa. Penso dunque che il Governo abbia la responsabilità

gli sia diano altre responsabilità e si mandi lì qualcuno che ci può andare. Non aggiungo altro, perché abbiamo scoperto quello che sapevamo, ovvero che con la Francia ancora non c'è un *dossier* completo, neanche in preparazione della nostra Conferenza di Palermo, alla quale verranno tutti.

hanno messo questo *dossier* in fondo, tra le carte ammuffite del Dipartimento di Stato, perché hanno altre priorità. D'altra parte, vedendo la politica di Trump, non ci si può meravigliare che la Libia non sia una priorità e questo rende ancora più difficile la nostra posizione. C'è da preoccuparsi:

Presidente, colleghi e signor Vice Ministro? Perché dopo sette anni dallo sciagurato intervento e dalla guerra in Libia, che - vorrei ricordare qui - fu decisa per ragioni che nulla avevano a che fare con l'ansia democratica di deporre un dittatore, purtroppo - ahimè - di crisi in crisi nessun passo avanti è stato fatto verso una speranza e un processo vero di stabilizzazione. Anche la tregua raggiunta grazie anche alla mediazione dell'ONU, come sappiamo, è fragilissima ed è stata violata ripetute volte; quella conclusa a Tripoli mercoledì scorso lo è ancora di più.

Tra l'altro, pochi giorni fa l'inviato dell'ONU Ghassan Salamé ha detto chiaramente - l'ha confermato anche il Ministro - che potrebbe non essere possibile tenere le elezioni nella data fissata,

quindi in contrasto con il Governo di Tripoli, e sarebbero comunque destinate a non risolvere nulla: potrebbero soltanto perpetuare la faida tra le due fazioni principali lasciando - questo è il problema della Libia - il territorio completamente in mano alle milizie armate che lo controllano, spesso senza riconoscersi nell'uno o nell'altro dei due fronti principali. Per gli interessi del nostro Paese - e ora mi soffermo sull'interesse dell'Italia - nulla, come abbiamo visto in questi sette anni, è più pericoloso di questa instabilità,

economici in campo energetico - sulle politiche dell'immigrazione e - su questo tornerò - con la lesione continua e costante dei diritti umani che avviene in Libia. Il nostro interesse, come Italia oltre che come donne e uomini che amano la pace, è riportare la stabilità in Libia: raggiungere il disarmo multilaterale delle milizie per arrivare a un vero e proprio patto tra tutte le forze in campo.

poter dialogare e stringere accordi in un ambito di riconoscimento e di costituzione di uno Stato. A ostacolare questo processo di pace purtroppo sono le stesse logiche che hanno provocato la destabilizzazione sette anni fa: la contrapposizione tra interessi di diversi Paesi europei che soffiano sul fuoco alla ricerca esclusiva dei propri vantaggi. Queste logiche ispirano ovviamente la forzatura di Haftar sorretta dalla Francia sulle elezioni di dicembre, ma io metto in guardia anche circa la Conferenza che si terrà che si terrà a Palermo il 12 e il 13 novembre, perché a mio avviso c'è il forte rischio, anche se gestita con maggior prudenza e minor avventurismo, che anch'essa finisca in un nulla di fatto.

spingere ancor di più, perché non sarà appoggiando una parte contro l'altra che si uscirà dalla tragedia in Libia, ma solo e unicamente rafforzando l'azione dell'ONU. Qui c'è una grande assente, ancora una volta dispiace dirlo,

peraltro più volte codificato in quest'Aula e in Commissione e dal lungo elenco delle attività svolte in queste settimane, per recuperare il terreno perduto. indubbio, infatti, che l'Italia è rimasta spiazzata da due eventi. Il primo è la Conferenza indetta in modo inappropriato dalla Francia mentre l'Italia era priva di un Governo:

di cui ancora non è chiara la motivazione, che hanno rischiato di mettere totalmente fuori gioco il nostro Paese. Di fronte a questi due eventi bene ha fatto il ministro Moavero con una serie di incontri internazionali (e noi ci auguriamo, essendo un partito patriottico, che si riesca nell'obiettivo), innanzitutto modificando la linea politica del nostro Paese con l'incontro con il generale Haftar (che non è una cosa casuale, ma è una modifica sostanziale della politica italiana nei confronti dei vari *partner* libici) e coinvolgendo anche l'altro attore che si era sentito escluso dalla nostra azione. Noi gli diamo atto che questa è stata una scelta saggia, non solo necessaria. Gli diamo inoltre atto di aver coinvolto tutti i soggetti possibili

nella convocazione di questa Conferenza per la Libia, cui però partecipano - lo diceva prima il senatore Casini in maniera appropriata - molti, troppi contendenti o partecipanti. Quando i partecipanti sono troppi, è anche difficile poi trovare un'intesa: la moltitudine fa emergere la debolezza. Il nodo di fondo è indubbio ed è ormai riconosciuto da tutti e noi siamo contenti che oggi tutte le parti politiche in questo Parlamento - mi auguro anche chi prenderà la parola subito dopo - faccia chiarezza su un punto:

e poi ripetutamente in questi sette anni (l'ultima volta appunto nel maggio scorso) contro gli interessi italiani, contro gli interessi libici (scatenando quello che ha scatenato) e contro gli interessi dell'Europa.

il Ministro degli esteri europeo, la signora Mogherini, faccia sentire la sua voce, tanto più in questo contesto, in cui gli interessi dell'Europa e gli interessi dell'Italia non sembrano convergere con quelli di un Paese europeo che si muove in sprezzo degli interessi generali e di quelli del nostro Paese. Per questo crediamo che sia importante in queste settimane, prima della Conferenza per la Libia, che si chiarisca questo aspetto. Il fatto di aver chiarito qui nel Parlamento nazionale e di avere oggi, a differenza di sette anni fa e anche di qualche tempo fa, la stessa sensazione nei confronti del contendente

tanto più laddove gli interessi strategici del Paese sono minacciati ripetutamente, come è stato conclamato in questi anni. Nella politica estera condivisa

Il Governo ha qualche settimana di tempo per chiarire con la Francia quale debba essere la posizione europea. Con riferimento a ciò, l'Unione europea deve necessariamente farsi sentire. Mentre

perché l'obiettivo è molto importante, l'Italia si espone molto e in quel teatro non possiamo perdere ulteriori colpi. Per questo chiediamo al Governo che si impegni realmente in queste settimane sul nodo di fondo. Non è la Russia, l'Egitto, il Qatar, l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, il Canada, la Germania, ma la Francia. Questo chiarimento deve essere fatto affinché la Conferenza abbia successo e l'Italia possa riprendere il proprio ruolo rispettato nel Mediterraneo.

di violenza e di vera e propria guerra civile. L'attacco della Settima brigata di Tarhuna è però il sintomo di una malattia più profonda che affonda le proprie origini nel mancato accordo sulla divisione sulla divisione delle risorse energetiche e sul controllo del territorio. In ultima analisi, direi che manca l'elemento essenziale della statualità, cioè il monopolio dell'utilizzo della forza. Dobbiamo partire da lì perché, se non si affronta quel tema, possiamo organizzare tutte le conferenze che vogliamo ma non otterremo mai un risultato duraturo. Mi ha allora soddisfatto solo in parte l'elenco degli invitati alla Conferenza del Ministro, che peraltro avevamo già sentito: non si è soffermato sulle criticità - salvo le parole che sottolineava il presidente Casini - e sulle difficoltà con la Francia. Deve dire con grande chiarezza quali sono gli obiettivi, con quali azioni e quali strumenti. Lo dico perché la Francia ha giocato le sue carte e insiste ancora per la data del 10 dicembre;

ma contano fra le proprie file l'ex funzionaria dell'ambasciata a Tripoli, adesso nominata vice rappresentante delle Nazioni Unite in Libia, che presenta un piano che nulla ha a che fare con il piano presentato da Salamé. Questa è la prima criticità evidente nelle parole del ministro Moavero Milanesi: dobbiamo sostenere Salamé, ma la sua vice rappresentante parla di un piano B che non prevede neanche il *referendum* costituzionale, ma delle elezioni parlamentari con la legge elettorale attuale, per poi addirittura annullare la risoluzione che prevedeva la legittimità delle istituzioni libiche. Insomma c'è molta confusione perché non sia solo una Conferenza in cui prevalgono la retorica e la celebrazione di un rito ma sia qualcosa di efficace, noi dobbiamo andare al cuore del problema e, affinché poi affinché poi in Parlamento ci si possa evidentemente trovare, il cuore del problema è il riconoscimento delle forze in campo, un riconoscimento politico alle milizie. Bisogna provare a mettere in campo un programma di vero e proprio disarmo, smobilitazione e reintegrazione, come è stato fatto in altri Paesi; se non si affronta il tema del controllo del territorio, del riconoscimento politico di chi lo controlla, noi mettiamo in campo delle conferenze che rischiano di essere un luogo in cui ci si parla solo addosso. Questo è il punto fondamentale di partenza e va fatto mettendo insieme gli attori principali, a partire dalla Francia, dagli Stati Uniti e dall'Unione europea. Questo vale per il controllo del territorio interno e anche esterno. Pensiamo al Niger, che è sottoposto a delle pressioni su più fronti: Boko Haram, dalla Nigeria, attraverso il lago Ciad, entra in Niger, la stessa cosa dal Mali con la presenza di Al Qaeda, per non parlare della crescita dei gruppi salafiti

vuole andare avanti, vuole anche rivedere le regole di ingaggio, ma è stato fatto un investimento. In questo momento noi in Niger non ci siamo e anche in questo caso con la Francia va trovato un punto d'accordo, a proposito di strumenti.

dei Paesi occidentali e l'Italia non c'era perché non era presente l'ambasciatore Perrone. È quindi necessaria la piena funzionalità della nostra ambasciata; inoltre, insieme a questo io direi di evitare che esponenti del Governo alimentino voci su presunte sostituzioni dei vertici dei nostri servizi di sicurezza perché da questo punto di vista noi rischiamo grosso. La credibilità dei nostri servizi di sicurezza è fondamentale in un'area come quella. permettetemi di fare una battuta sulla cooperazione con la Libia sui flussi migratori. Nel luglio 2017, sotto la spinta del governo Gentiloni Silveri, ci siamo mossi su due versanti: accordo con le tribù per fermare la tratta degli esseri umani e i flussi migratori e, dall'altra, l'apertura dei centri di permanenza aprendo al controllo delle organizzazioni internazionali. Oggi il nuovo Governo arretra, si ritira, porta indietro i dispositivi di sicurezza del nostro Paese; si allarga l'area *search and rescue* (SAR) libica con una deterrenza non solo nei confronti delle organizzazioni non governative, ma anche nei confronti delle navi di Frontex, finanche (come abbiamo visto nel caso della nave Diciotti) nei confronti della Guardia costiera libica.

Si sta assottigliando quella linea sottile - lo diciamo con tutta la moderazione del caso - tra l'essere uomo di Stato a tutela delle linee tradizionali della politica estera del nostro Paese e l'essere invece la foglia di fico di politiche che portano qualche *like* in più su Facebook, ma ci isolano nella comunità internazionale, con gravi rischi per la stabilità e la sicurezza del nostro Paese.

innanzitutto vorrei ringraziare il Ministro per la disponibilità che ha dimostrato fino ad ora e che sta confermando nell'informativa rispetto alla questione della Libia; disponibilità che ha palesato sia oggi in Aula, sia con le audizioni nelle Commissioni che hanno dato modo a noi membri del Parlamento di svolgere la nostra funzione. La situazione che ci ha descritto oggi e nel recente passato certamente porta a sviluppare molte riflessioni che devono portare, con il confronto interno, a concorrere a determinare la linea che l'Italia deve avere nelle relazioni con lo scenario libico; ciò, ovviamente, prescindendo da facili strumentalizzazioni politiche interne. La situazione di instabilità politica libica, così come ci viene confermata anche dalle agenzie che si susseguono giorno per giorno, deve essere assolutamente ricondotta a canoni ordinari, così da permettere un'altrettanto ordinaria disamina delle problematiche interne ed estere. Da un lato la questione libica, com'è stato opportunamente delineato, non può essere affrontata senza un rafforzamento della posizione italiana tale da fungere, secondo gli usi della diplomazia, come agente proattivo per il componimento bonario delle reciproche pretese. Sul punto oggi il Ministro ci ha rassicurato, rassicurato, confermando la Conferenza di Palermo che, a differenza di quanto detto da altri, riteniamo un punto importante, fondamentale perché quello sì, è stato un momento di scambio reale per cercare arrivare ad una soluzione concreta. Dall'altro, non possiamo tacere come le influenze estere, al di fuori dei richiamati tavoli diplomatici, debbano essere limitate o comunque coordinate con il rafforzamento dell'opera delle Nazioni Unite, così da consentire davvero un consolidamento di quegli equilibri interni e quindi dare finalmente stabilità a tutto il Paese. In tale quadro generale occorre sottolineare e ricordare come lo stallo di questa situazione, che rischia di protrarsi ulteriormente, altro non fa che mettere a repentaglio, come confermato dal Ministro anche oggi, le calendarizzate elezioni interne che, secondo un processo democratico, dovrebbero portare alla definitiva stabilizzazione interna. Sappiamo che questo percorso, così come stabilito al vertice di Parigi del 29 maggio, oggi sia in pericolo. Ce lo ha confermato oggi il Ministro. In tale quadro generale occorre sottolineare che in questo stallo abbiamo l'obbligo di provare a portare ordine ove questo manchi secondo i compiti e i ruoli internazionali. In questo quadro le strumentalizzazioni politiche interne dovrebbero venire meno, strumentalizzazioni politiche da parte delle opposizioni che spesso richiamano a soluzioni fumose e idealiste che tutelino, sì, il rispetto dei diritti umani ma che da un punto di vista pragmatico sono solo palliativi e non fanno altro che alimentare le tensioni. Oggi dobbiamo renderci conto che strumentalizzare la questione libica al solo fine di giustificare l'incondizionata e ingiustificata tratta di esseri umani verso il nostro Paese, è idea profondamente sbagliata, sbagliata, in primo luogo per le popolazioni che arrivano dal continente africano. Da questo punto di vista bene fa il ministro Moavero Milanesi a sottolineare la discussione di confronto, come ha ribadito in passato durante le audizioni, con tutto il collegio dei Ministri, affinché si possano condividere idee e soluzioni. Non posso peraltro sottacere come anche nelle audizioni vi siano stati attacchi a nostro dire palesemente ingiustificati e assolutamente provocatori da parte di esponenti delle minoranze con il solo recondito scopo di ribadire una strumentale posizione contraria alla politica del Governo. Forse, però, in questa discussione dobbiamo resettare tutto. Proviamo a ripartire da semplici concetti e obiettivi chiari, così da poter comprendere e focalizzare il traguardo che il Governo italiano deve perseguire e raggiungere. *In primis* dobbiamo adoperarci affinché il lavoro diplomatico sia realmente produttivo e consenta concretamente il componimento degli scontri libici, così che l'instabilità cessi, perché questo è il concetto di base. Se riusciamo a dare stabilità ad un Paese, riusciamo anche ad aiutare la popolazione in questo stesso Paese e se riusciamo ad aiutarlo mediante strutture organizzate, efficaci e trasparenti, abbiamo raggiunto il risultato di far rispettare quei diritti umani che oggi vengono utilizzati solo come pretesto per alimentare uno sporco mercato ed una tratta L-SP-PSd'Az)*. Ma forse pensiamo che giustificare l'instabilità politica libica mediante un'accoglienza incondizionata sia la soluzione? No, davvero non lo crediamo. Non possiamo pensare di giustificare l'immigrazione clandestina in Italia e in tutta Europa dicendo che serve per salvare vite umane. Noi abbiamo invece l'imperativo categorico, se non morale, di portare aiuto senza creare un male più grande di quello che vogliamo curare. Abbiamo già visto come nel recente passato gli interventi unilaterali cosiddetti umanitari, messi in atto con le forze armate da parte di taluni *partner* europei, abbiano nel concreto aggravato la situazione, creando solo ulteriori ingiustizie e negazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Pensiamo davvero che la diplomazia possa essere utile a corrente alternata? Oggi lo Stato italiano si trova a dover svolgere, anche per colpe di altri, un compito molto difficile, che però potrebbe essere molto più agevole ove vi fosse una maggiore incisività da parte dell'Europa nella politica estera. Ciò, però, tarda a pervenire. Ove questa manca, ecco che allora noi dobbiamo farci carico dell'onere di facilitare una stabilizzazione della Libia. Questo lo dobbiamo innanzitutto per il rispetto delle vite umane che vogliamo salvaguardare, affinché coloro che oggi divengono - forzosamente e forzatamente possano essere liberi cittadini, ognuno nel proprio Paese e nella propria Nazione. Egregio Presidente, prima di intervenire vorrei rivolgerle una mozione degli affetti parlamentari. Siamo grati al sempre cortese ministro Moavero Milanesi della sua presenza, ma siamo qua non solo per ascoltare, ma anche per essere ascoltati. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Forza Italia vigila e sempre vigilerà perché non venga svuotata questa istituzione, che è uno dei cardini della nostra democrazia. Capisco le esigenze del Governo, ma mi auguro che una simile mancanza di garbo istituzionale non si ripeta più. Grazie, signor Presidente. È del tutto superfluo ribadire l'importanza che la partita libica riveste per il nostro Paese e per l'area mediterranea tutta. Lo è non solo per la questione migratoria, che sta a cuore a tutti noi, ma anche e soprattutto

che si deve caratterizzare, differentemente dagli ultimi anni e dagli altri *partner* europei, come forza di pace, dialogo e sviluppo condiviso nell'area euro-mediterranea. Quanto accaduto e accade in queste ore in Libia, che - non dimentichiamolo mai - è una delle porte sull'Africa, è la dimostrazione di come serva, oggi più che mai, un'Europa politica e una politica estera europea, che saranno non gli attacchi all'Unione europea a costruire, ma un progetto di cui il Governo sembra non curarsi. Se non ci chiariremo tra *partner* europei - *in primis*, noi e la Francia difficilmente verremo a capo di questa partita e condanneremo la Libia e tutta l'area a una lunga stagione di caos. Consideriamo questo necessario, perché è difficile teorizzare, anche con tutta la retorica in possesso di questo Governo, che la Libia rientri oggi tra gli interessi strategici dell'America trumpiana. Del resto, nonostante gli annunci *spot* del presidente Conte, non si è ancora neanche capito se il Trump sarà presente alla Conferenza sulla Libia. sono la riprova delle storture e degli errori che hanno caratterizzato il processo di pace libico e la creazione di un'entità statuale: errori - dobbiamo dircelo con sincerità - a cui, come Paese, non siamo estranei. Sebbene consideriamo uno sbaglio celebrare in Libia elezioni il 10 dicembre prossimo, come prefigurato sotto dettatura lo scorso maggio a Parigi e come peraltro dichiarato anche ieri dall'inviato ONU in Libia Salamé, consideriamo altrettanto rischiosa, specie sulla scorta delle esperienze recenti, ogni scelta e iniziativa che possa far apparire il nostro Paese un attore di parte, non terzo, tra le fazioni in campo. È un errore che abbiamo già commesso in passato, dopo la caduta di Gheddafi, e che non ha fatto le fortune nostre, né della Libia. Per questo motivo, abbiamo apprezzato il tentativo del ministro Moavero Milanesi di avviare un dialogo con il generale Haftar. Tale apprezzamento non può però riguardare i silenzi del Governo sulle richieste delle tribù del Sud, dai Tebu agli Awlad Suleiman, passando per i Tuareg. Eppure, i Tuareg libici, per bocca del *leader* Moulay Kamidi, hanno chiesto al Governo italiano di offrire aiuti concreti alla realtà del Sud. Al pari, ci sono accuse recentissime, mosse da tutte le tribù del Sud al nostro Governo e al Governo libico da noi sostenuto, di mancanza di serietà e sincerità nell'applicazione dell'accordo sottoscritto a Roma nel maggio del 2017. Davanti a queste richieste l'Italia è rimasta silente. Ma il Sud libico è per noi strategico. È l'area da dove giungono i flussi di migranti, dove si giocano importanti partite energetiche e dove la situazione oggi è molto grave, in particolare a Sebha,

al fine di aver chiari i nostri interessi, il nostro ruolo e la direzione che, come Italia, dobbiamo intraprendere, specie in vista della Conferenza internazionale sulla Libia prevista per metà novembre a Palermo, che il Governo intende promuovere. È un'iniziativa di cui è necessario definire i contorni e gli obiettivi; il ministro Moavero Milanesi oggi non ce li ha spiegati. Abbiamo letto tutti in questi giorni le indiscrezioni che parlano delle condizioni che il generale Haftar avrebbe posto per partecipare alla Conferenza. Non vorremmo però che, per avere a quel tavolo Haftar, che abbiamo lungamente non riconosciuto, magari per una bella foto *opportunity*, accondiscendessimo a tutte le sue richieste, alcune rischiose - penso all'assenza di gruppi a Tripoli (che potrebbe favorire una invasione militare)

pertanto chiarezza, ma a tal fine non aiutano le posizioni di alcuni membri del Governo, che escludono *a priori* qualsiasi nostra presenza militare in Libia (peraltro in Libia i militari italiani già ci sono), specie dopo la richiesta di ieri di Tripoli all'ONU. In Libia la forza militare conta e tante milizie sono pronte a mettersi con il più forte, anche se non possiamo pensare di rafforzare una posizione debole, come appare quella di Sarraj, con il solo impiego della forza. La strada è quindi stretta. Ma al tavolo della Conferenza, allo stato assai fumoso, serve uno sforzo di condivisione e di dialogo, che interessi con franchezza, oltre che le parti libiche, anche gli altri attori europei (in tal senso ha ragione il Ministro degli Gli annali sono pieni di conferenze inutili; dobbiamo lavorare per non aggiungerne un'altra. *(Applausi

io credo che anche oggi abbiamo assistito a una pagina nuova nella politica italiana, perché il ministro Moavero dato seguito a quelle che sono state le nostre richieste in altre situazioni e ha prontamente dato la sua disponibilità a venire a riferire in Aula, a nostro modo di vedere su molte novità dello scenario libico. questo è soltanto uno degli ultimi atti del Governo del cambiamento, di cui vorrei sottolineare alcuni aspetti. Uno, in particolare, secondo me è fondamentale: mi riferisco al fatto che il Governo italiano stia

eventi che sono stati portati avanti dal nostro Governo. Il 29 agosto il nostro vice *premier* Di Maio è stato in visita in Egitto. All'inizio di settembre - come abbiamo ascoltato - il ministro Moavero Milanesi è stato direttamente in Libia, a Bengasi, per interloquire con il generale Haftar. La scorsa settimana, durante l'Assemblea generale dell'ONU, il nostro *premier* Conte ha avuto una serie di incontri bilaterali con lo stesso al-Sisi sulla situazione egiziana. Il ministro Salvini è stato ripetutamente sui territori sui territori africani, non da ultimo quello tunisino. Questo dimostra sostanzialmente un cambio di passo fondamentale del Governo italiano, grazie proprio al Governo del cambiamento, perché mai si era visto un attacco frontale istituzionale verso una problematica di questo tipo; cosa sicuramente che non era accaduta negli scorsi anni.

per la situazione e la stabilità democratica anche del nostro Paese. È chiaro che, come ha riportato il ministro Moavero Milanesi, la situazione in Libia è tutt'altro

di pace di Palermo che, giustamente, il Ministro ha chiesto di svolgere non nella nostra capitale, che è sede di tante istituzioni importanti, ma proprio nella Regione che è la nostra frontiera verso quello scenario. Credo che questo sia un dato estremamente importante. Qualcuno ha chiesto quali fossero le novità; signori, le novità sono queste: mai in otto anni era stata convocata una Conferenza di pace sulla Libia e lo stiamo facendo noi, chiamando gli attori principali di questo scenario. Questo sicuramente non farà altro che rinforzare la nostra «egemonia» su una determinata area, che sicuramente porterà benefici non soltanto a noi, ma anche in quei territori. Spero, dalle notizie che arrivano dal terreno, che possa essere coinvolta in qualche misura anche la Giordania. Vedo

Democratico, non ho bisogno di leggerla perché credo fermamente nelle parole che dico e quindi non ho bisogno di leggere la frasetta che mi è stata preparata. Credo che il Governo del cambiamento passa anche da qui, attraverso un nuovo modo di fare politica estera.

fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018;* b) *Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti,

l'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati recante ratifica ed esecuzione dei Trattati e del relativo scambio di note, sottoscritti dall'Italia e dagli Emirati Arabi Uniti a partire dal settembre 2015, rispettivamente in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale. I due accordi bilaterali rientrano nell'ambito di quell'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria internazionale con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea,

mediante una più stretta collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione e dell'assistenza giudiziaria in materia penale. Il primo dei due Trattati in esame, quello in materia di estradizione, fatto ad Abu Dhabi nel settembre 2015, integrato da uno scambio di note il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018, e composto da 24 articoli, è finalizzato a consentire l'estradizione obbligatoria, secondo le norme e le condizioni indicate, di persone ricercate che si trovino nel territorio di uno dei due Paesi per dare corso a un processo penale o al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva. Il testo prevede che l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il principio della «doppia incriminazione». Tale principio trova tuttavia un temperamento in materia fiscale, laddove viene previsto che l'estradizione possa essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente. L'estradizione processuale richiede, inoltre, che il reato per cui si proceda sia punito da entrambi gli Stati con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda a un periodo minimo di sei mesi. Il testo disciplina altresì i motivi obbligatori per opporre un rifiuto all'estradizione, prevedendo, fra l'altro, oltre ai casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quelli relativi a reati puniti dallo Stato richiedente con pene proibite dalla legge dello Stato richiesto, o quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a tortura o a trattamenti illegali e disumani. Viene inoltre previsto un rifiuto obbligatorio anche nel caso in cui il reato per il quale venga chiesta l'estradizione sia punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato richiedente, salvi i casi in cui la pena capitale non sia inflitta nei confronti della persona richiesta, ovvero, qualora già inflitta, lo Stato richiedente assuma l'impegno di non darvi esecuzione. A tal riguardo lo scambio di note fra i due Paesi risalente al novembre 2017 e al gennaio 2018 ed allegato al Trattato, prevede, conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, che resti esclusa del tutto la possibilità di dare luogo a estradizione nei casi in cui sia prevista la pena di morte, a meno che la parte richiedente non adotti una decisione irrevocabile che commuti tale pena in una pena diversa, nel pieno rispetto dell'ordinamento della parte richiesta. Il Trattato indica inoltre i motivi facoltativi per opporre un rifiuto all'estradizione, riferibili ai casi in cui lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione o abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, o a valutazioni di carattere umanitario in relazione all'età e alle condizioni di salute della persona da consegnare. Il testo, dopo aver individuato nei rispettivi Ministeri della giustizia le autorità centrali preposte all'attuazione del Trattato, disciplina le modalità e i documenti necessari per la presentazione di una richiesta di estradizione, pone un generale divieto di riestradizione della persona consegnata, fissa le procedure per la consegna della persona e stabilisce che la composizione delle controversie interpretative o applicative fra le parti avvenga mediante consultazione in via diplomatica. diplomatica. Il secondo Trattato oggetto del presente disegno di legge di ratifica - quello relativo alla mutua assistenza giudiziaria in materia penale - si compone di 25 articoli ed è finalizzato a disciplinare l'assistenza giudiziaria penale bilaterale. L'adozione di tali norme è stata imposta dalla progressiva estensione dei rapporti economici, commerciali e finanziari tra i due Paesi, aspetto che inevitabilmente reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che rendono necessaria la predisposizione di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione bilaterale. Il testo esplicita l'impegno delle parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale - ed espressamente anche in relazione a reati tributari e fiscali prevedendo fra l'altro la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti ed elementi di prova e di informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'effettuazione di attività di indagine, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose a esso pertinenti. Il Trattato, che prevede anche lo scambio di informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini, nonché la possibilità di dar luogo a qualsiasi forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto, disciplina quindi le modalità per la formulazione delle domande di assistenza, nonché i casi per l'opposizione di un rifiuto a tali richieste. Di particolare rilievo, a tal proposito, Di particolare rilievo, a tal proposito, la previsione secondo cui l'assistenza non possa essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie, ovvero in ragione del fatto che il reato si consideri anche di natura fiscale. Ulteriori articoli definiscono le modalità per l'esecuzione della domanda, per la notifica degli atti, per l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, per il transito di persone in stato di detenzione, per l'effettuazione di perquisizioni e sequestri relativi a una procedura penale. Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore. Gli oneri economici per l'Italia derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati in 40.000 euro annui, a decorrere dal 2018. I due Trattati in esame non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

*(PD)*. Signor Presidente, cari colleghi, il provvedimento in esame riguarda due Trattati tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti in materia giudiziaria. I due Trattati si inseriscono nel contesto degli strumenti finalizzati alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione fra l'Italia e Paesi non appartenenti all'Unione europea, allo scopo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto alla criminalità. In questo caso, viene avviato un processo di sviluppo significativo dei rapporti italo-emiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Paesi in ogni settore: dall'economia al mondo della finanza, al commercio, ai flussi migratori. II progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali, che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente le procedure di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono scontare una pena e l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione. Gli accordi rientrano in un percorso di cooperazione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, che riguarda vari settori: come ho detto prima, dall'ambito finanziario all'economia, al turismo, alla cultura. Era ed è necessario aggiungere questo tassello della cooperazione giuridica in tema di estradizione e, quindi, a contrasto della criminalità transnazionale. È un percorso che ci permette di disciplinare e rendere più fluide le procedure di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire e scontare una pena. Ad oggi, 14 casi di italiani latitanti di fatto negli Emirati Arabi Uniti, che con questo provvedimento potranno essere estradati e riportati in Patria...

Stavo dicendo che, ad oggi, 14 casi di italiani latitanti, di fatto, negli Emirati Arabi Uniti, che con questo provvedimento potranno essere estradati, riportati in Patria e assicurati, quindi, alla giustizia italiana, mettendo fine ad un fenomeno che ha giustamente creato e suscitato stupore e sdegno nella nostra comunità, cioè che i responsabili di crimini non avrebbero mai pagato la pena. Credo che oggi stiamo attendendo ad uno dei nostri doveri da eletti del popolo. Ristabiliamo i principi di legalità e di giustizia e permettiamo anche alle nostre aziende che vanno in quei Paesi la certezza del diritto, che è alla base di qualunque sviluppo pacifico, di qualunque tipo di relazione. Signor Presidente, noi del Partito Democratico sosteniamo questo provvedimento, non solo perché anche noi l'abbiamo presentato, non solo perché è il frutto di un lavoro dei Governi a guida Renzi e poi Gentiloni Silveri, ma anche perché si tratta di un atto importante contro la criminalità e le mafie. È un provvedimento che si colloca nel solco di altri provvedimenti importanti della passata legislatura: dalla legge contro il caporalato, alle leggi per istituire il reato di antiriciclaggio, per inasprire il voto di scambio politico-mafioso, per combattere i reati ambientali. Per questo, dunque, la ratifica, secondo noi, è molto importante, non solo per assicurare alla giustizia italiana delle figure che sono fuggite, ma anche come elemento di deterrenza, perché si afferma che non c'è più, a poche ore di volo, un'oasi di latitanza; non c'è più la possibilità di farla franca. Concludo, signor Presidente, con l'auspicio che questo provvedimento possa essere approvato con il più ampio voto del Senato.

scontare la pena, penso sia qualcosa di giusto, equo e importante per il nostro Paese. È interessante il punto sulla reciprocità.

colleghi e colleghe, finalmente, dopo anni, giunge in quest'Assemblea il testo finale del provvedimento che regola i rapporti tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti in materia di assistenza giudiziaria penale ed estradizione tra i due Governi.

Un accordo che, per quanto riguarda l'estradizione di cittadini arrestati o destinatari di un processo nei Paesi d'origine, stabilisce un principio molto importante:

in Paesi di orientamento diverso per quanto riguarda l'espiazione della pena. Un primo passo importante, ma bisogna certo fare di più. Immagino nel futuro una piattaforma normativa in cui alcuni reati tipici del nostro Paese possano essere riconosciuti dai firmatari di accordi per l'assistenza giudiziaria penale. Immagino il 416-*bis*, che sia universalmente riconosciuto come reato da tutti i Paesi del mondo, anche perché ormai considerare la mafia come organizzazione criminale nazionale è antistorico e, se posso permettetemi, anche irresponsabile. La riprova, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ce la può fornire la Germania, che qualche anno fa ebbe una sanguinosa guerra di 'ndrangheta, ricordata come strage di Duisburg, oppure la Gran Bretagna, con la colonia di latitanti italiani che riciclano denaro della mafia nella *City*, per non citare la Spagna o alcuni Paesi dell'Est Europa. Ad ogni modo, un passo importante è stato fatto. La ratifica di questo accordo deve essere prodromica per rilanciare un progetto di rapporti giudiziari con altri Paesi non sottoscrittori, quasi tutti definiti paradisi fiscali. Ricordo infatti che gli Emirati arabi non hanno sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'estradizione, che è stata firmata a Parigi nel 1957. Dobbiamo rendere difficile ai criminali spostarsi e trovare rifugio in altri Paesi. Per chiarezza, bisogna sottolineare che, anche dopo la ratifica, il Trattato in questione non potrà regolare che le procedure di estradizione attivate dopo la sua entrata in vigore, ma è chiaro che per l'estradizione dei latitanti dimoranti nel Golfo sarà cura del Ministero della giustizia attivarla già dal giorno successivo all'approvazione dell'Assemblea della citata ratifica del Trattato. Naturalmente questo Trattato va ad intendersi in un rapporto più ampio, che tocca temi di carattere economico, finanziario e del turismo e una puntuale sottoscrizione non può che rendere più agevoli i già importanti rapporti

Signor Presidente, vorrei chiedere l'attenzione dei colleghi, perché l'argomento di cui sto per parlare non penso ci riguardi come rappresentanti di partiti politici, ma come persone ed esseri umani. È con tristezza, cari colleghi e signor Presidente, che intervengo per parlare della tragedia in Indonesia, uno dei Paese della mia ripartizione elettorale. contano oltre 1.200 vittime, a causa del violento terremoto di magnitudo 7.4 e del conseguente tsunami, una tragedia che si ripete dopo quella del 2004 e il devastante tsunami a Sumatra. Purtroppo il numero delle vittime è destinato a salire. Molte sono le persone ancora sotto le macerie, molte sono le aree da raggiungere e nuove scosse di terremoto si ripetono, anche in altre isole dell'Arcipelago indonesiano: di qualche ora fa la notizia di una scossa di magnitudo 5.9 nell'isola di Sumba. Le zone colpite sono molto estese e difficili da raggiungere: mancano quindi acqua e beni di prima necessità e c'è il rischio di epidemie. L'onda anomala dello *tsunami* ha colto di improvviso la popolazione di Palu e Donggala. Subito dopo il terremoto era stata diramata anche un'allerta, rientrata però dopo un'ora. All'improvviso, però, il muro d'acqua e le onde anomale alte oltre due metri si sono abbattuti con tutta la loro violenza sulla costa, causando morte e distruzioni. Purtroppo, come sappiamo, non è possibile prevedere un terremoto, ma una più attenta analisi, forse, avrebbe potuto evitare o limitare il disastro dello tsunami. È necessaria la collaborazione e la cooperazione tra gli organi internazionali per migliorare i sistemi di allerta per eventi come questo. Il dramma in Indonesia sta assumendo dimensioni enormi ed il Governo indonesiano ha chiesto aiuto ed assistenza alla comunità internazionale. Io spero che ci si possa impegnare tutti nell'aiuto a questa popolazione. Signora Presidente, certo di interpretare il sentimento di tutte le senatrici ed i senatori, permettetemi di concludere esprimendo il nostro dolore, il cordoglio e la nostra solidarietà al popolo indonesiano.

questione di proporzioni enormi, perché riguarda oltre 150.000 esercizi coinvolti (bar gastronomie, ristoranti, piccola e grande distribuzione), oltre 90.000 imprese che hanno acquistato questi

Della vicenda, come dicevo prima, ne avevamo parlato già a luglio, quando stava per esplodere la questione. Negli scorsi giorni, dopo il fallimento, c'è stato un allarme enorme sia per chi, aziende e cittadini, è rimasto in possesso di questi buoni pasto di cui ormai non si capisce più quale potrebbe essere l'utilizzo, sia per la sia per la situazione dei lavoratori colpiti da tale situazione. Il problema è che né il Ministero sembra in grado di dare una prospettiva, né la curatela e la proprietà stanno dando segnali di vita. In più, negli scorsi giorni si è palesata un'ulteriore situazione che ha del paradossale: Consip sembra aver assegnato

dei disastri che rischiano di ripercuotersi su imprese che hanno ricevuto in pagamento questi buoni e che adesso non sanno cosa farsene, su imprese che li avevano acquistati e se li sono ritrovati in carico, su singoli cittadini che li avevano ricevuti dalle imprese e che li hanno in mano, nonché sui lavoratori, questa rischia di essere una bomba veramente esplosiva. Chiediamo in modo accorato che il Ministero prenda in mano la situazione e che, se del caso (noi riteniamo proprio di sì), risponda alle nostre interrogazioni.

Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, il presente intervento è dettato dalla necessità di portare anche in quest'Aula un tema dibattuto nell'altra ala del Parlamento, che con 295 voti favorevoli e 181 contrari ha accettato le dimissioni del deputato Andrea Mura, già espulso dal nostro Gruppo parlamentare per avere totalizzato oltre il 96 per cento La grande eco mediatica ha contribuito a creare un vero e proprio caso sul quale si è registrato un elevatissimo numero di dichiarazioni da parte dei rappresentanti delle opposizioni, i quali hanno espresso inaccettabili, pesanti e vergognosi giudizi sull'operato del MoVimento 5 Stelle per aver scelto - secondo loro - un candidato sbagliato, guardandosi bene dall'andare oltre il caso Mura, come una matura riflessione politica avrebbe preteso, ed affrontare responsabilmente - ed aggiungo, finalmente - il problema dell'assenteismo dei parlamentari. Tutto ha preso le mosse dalla denuncia del deputato di Forza Italia Ugo Capellacci, ex Presidente della Regione Sardegna - che alle elezioni politiche del 4 marzo venne battuto nel collegio uninominale di Cagliari proprio da Andrea Mura - il quale, attingendo dai dati ufficiali della OpenParlamento, segnalava l'alto tasso di assenze del deputato Mura, anche componente della Commissione parlamentare trasporti, poste e telecomunicazioni. Alle risposte poco edificanti che non fornivano giustificazione alcuna da parte di Mura («L'attività parlamentare si può svolgere in barca», diceva), è seguito, come tutti sanno, l'intervento del MoVimento 5 che, come sempre, è stato lineare, attento a garantire il rispetto delle regole e l'applicazione dello statuto e del codice etico, ma soprattutto il rispetto della Costituzione della Repubblica e delle leggi. Da qui il consequenziale provvedimento di espulsione del signor Andrea Mura, il quale solo il 4 agosto annunciava le sue dimissioni da parlamentare con una lettera inviata al presidente della Camera Roberto Fico, nella quale, peraltro - spiace sottolinearlo - non vi è traccia minima di scuse per non aver ottemperato all'obbligo di presenziare ai lavori parlamentari come imposto dallo statuto, dal codice etico e dalla stessa funzione pubblica assunta. L'accettazione delle dimissioni da parte della Camera è storia recente e sarebbe il naturale epilogo di cui prendere atto senza ulteriori osservazioni, se non fosse per il numero davvero spropositato di dichiarazioni dell'opposizione e della loro portata contraddittoria che si può condensare nella frase: «Voi del MoVimento 5 Stelle non avete nulla da insegnare». Analizzando con lo stesso rigore i dati aggiornati, resi pubblici qualche giorno fa, si viene a sapere che il deputato più assenteista è la forzista Michela Vittoria Brambilla, alla sua quarta legislatura,

per la sua costituzione). Le stesse forze politiche che in modo offensivo e contraddittorio si sono rivolte al MoVimento 5 Stelle non accorgendosi della trave che è nel loro occhio, evidentemente oltre a non avere la stessa dirittura morale del MoVimento 5 Stelle, non ne hanno la linearità, il coraggio e la fermezza necessari per far rispettare le regole. Ecco perché si chiede un cambio di passo e si pretende che applichino lo stesso metro di giudizio nei confronti dei propri eletti ed i conseguenti provvedimenti anche in casa loro. Concludo, signor Presidente, nella speranza che l'assenteismo dei parlamentari diventi oggetto di riflessione seria e responsabile da parte di tutta la classe classe politica e che lo stesso Consiglio di Presidenza prenda in seria considerazione i casi segnalati con questo intervento. *(Applausi dal